dell'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato in relazione alla manovra di bilancio: egli ha accusato il Governo di falso ideologico. Poiché l'amministratore delegato è nominato dall'azionista con un rapporto fiduciario, delle due l'una: se ha ragione Moretti, il Governo deve prenderne atto e i Ministri interessati si devono dimettere. l'azionista, dunque il Governo, ha l'obbligo di togliere la fiducia all'amministratore delegato. Non è possibile che in questo Paese i *commis* dello Stato si alzino e dicano ciò che hanno in testa a ruota libera,

Questo parere lo revoco, perché vi è stata una non corretta interpretazione del testo. Quindi, sull'intero emendamento il parere è contrario,

pone a carico dei Comuni indistintamente la ripartizione dei risparmi, mentre invece la precisazione è che i risparmi vanno fatti gravare su quei Comuni nei quali si verifica l'anomalia. Quindi, non Quindi, non è una norma nuova in senso sostanziale, ma una mera precisazione del criterio di riparto di queste risorse, o meglio di questi tagli, perché di questo parliamo.

al fine di trovare perfetta e puntuale compensazione anche degli effetti complessivamente stimati dal disegno di legge all'attenzione e dai relativi emendamenti approvati dalla Commissione sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, che è stato nei giorni scorsi oggetto di dibattito, di attenzione e, infine, anche di un'apposita riunione della Commissione bilancio. Ebbene, l'emendamento 14.800

la frase riportata tra virgolette del comma 8 dell'articolo 14 che, sulla base di un emendamento a suo tempo approvato dalla Commissione, apportava una rettifica alle norme sul patto di stabilità interno per escludere dalle stesse le opere cofinanziate dall'Unione Europea, a partire dall'anno 2009. Con questa proposta emendativa verrebbe a cadere tale modifica, riportando il testo alla sua versione originaria, così come contenuta nel disegno di legge finanziaria approvato dal Consiglio dei ministri. La seconda parte, anch'essa tecnica, comporta una correzione dell'articolo 79 della norma con la quale si rendono più efficienti le operazioni di manutenzione degli immobili appartenenti al demanio dello Stato, per espungere da tale ambito di applicazione gli immobili detenuti da altri enti o organismi pubblici, così come individuati in un apposito elenco dell'ISTAT. Infine, e questo è il vero e proprio emendamento, con riferimento all'anno 2008, si riduce la Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 15 milioni di euro, e con riferimento alla Tabella C, sempre alla voce Ministero dell'economia e delle finanze - Fondi di riserva, si riduce l'importo per 82 milioni. Ovviamente, le correzioni apportate alla Tabella A A riguardano non solo la voce ora ricordata di 15 milioni, ma integrano la Tabella A per gli anni 2009-2010 di un importo pari a 313 milioni per anno, derivante dalle conseguenze apportate dalle due proposte tecniche che ho dinanzi ricordato. Quindi, l'effetto complessivo dell'emendamento è, in particolare, quello di individuare, sulla base delle migliori stime, una piena compensazione che l'insieme delle norme contenute nel disegno di legge finanziaria produrrebbero negli anni 2008, 2009 e 2010 sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, quindi recependo in pieno l'indicazione che è stata data dalla Commissione bilancio, la quale a sua volta ha anche recepito la discussione approfondita che si è tenuta in Aula.

il lavoro in Commissione ha integralmente sostituito il testo iniziale dell'articolo 14, acquisendo un tema per noi fondamentale, che è giusto tagliare i costi impropri della politica ma non è possibile, in nome di ciò, tagliare le articolazioni e le risorse della democrazia. Nel testo del Governo venivano tagliati oltre 20.000 consiglieri comunali e, in realtà, in questo modo si limitava la soglia d'accesso, dando un colpo alla rappresentanza democratica delle minoranze. Al contrario, e noi perciò siamo d'accordo, l'emendamento approvato in Commissione e redatto dal relatore, certamente incide sui costi, il che è positivo, ma salva l'articolazione democratica. Il mio Gruppo, tuttavia, ha una preoccupazione e la riflessione che voglio fare è proprio questa: perché il Governo è arrivato

ma, ovviamente, qui ed oggi, bisogna vedere come è possibile ridurre i costi impropri della politica, che per nostra iniziativa sono stati ridotti anche con altri importanti emendamenti, per esempio quello che riguarda i tetti stipendiali. Il tema è quello di evitare abusi, fare più commissioni di quelle che realmente si fanno, sedute, vincoli e questo è ben presente nel lavoro svolto in Commissione. Ci è sembrato anche giusto eliminare l'aspettativa per incarichi consiliari e non amministrativi. Avremmo però preferito, forse è una svista, che l'aspettativa fosse mantenuta per i Presidenti delle circoscrizioni o municipalità delle grandi città metropolitane. Infatti, il Presidente di Cinecittà a Roma o di Scampia a Napoli è Presidente di un territorio che rappresenta una comunità di oltre 100‑150.000 persone, ed è inoltre importante che si sia difesa l'articolazione delle circoscrizioni sotto i 100.000 abitanti, rendendole a presenza volontaria. Credo, quindi, da questo punto di vista, che sia giusto votare. Vogliamo segnalare che certamente, data la fretta con cui è stato svolto questo buon lavoro per risolvere il delicato problema posto dal Governo che a nostro avviso, lo ripeto ancora, era più un taglio della democrazia che dei costi, si potrebbe affrontare qualche problema tecnico che potrà essere corretto, magari in fase successiva, con la stessa riforma delle autonomie. Inoltre, vorremmo porre un ulteriore tema di riflessione: noi siamo noi siamo favorevoli che le competenze dei Consigli comunali siano valorizzate e vogliamo evitare che tutto si riduca, negli enti locali, a dare più potere ai Sindaci e alle Giunte. Per questo siamo stati d'accordo con la riduzione dei componenti delle Giunte delle città metropolitane, quando saranno finiti i mandati, e saremo sempre d'accordo, al di là dell'aspetto delle indennità e delle retribuzioni, a dare centralità al ruolo dei Consigli che sono diretta espressione della democrazia e che svolgono un ruolo di indirizzo e di controllo.

però - lo ripetiamo ancora - in una funzione che eviti che in nome dei costi qualcuno riduca la democrazia e concentri il potere negli esecutivi e nei sindaci.

abbiamo 790 consigli di circoscrizione, con 12.541 consiglieri,

abitanti); Guidonia, con 68.000 abitanti, 9 circoscrizioni e 144 consiglieri (1 ogni 450 abitanti); abitanti); Gorizia, con 35.000 abitanti, 10 circoscrizioni, 132 consiglieri (1 ogni 260 abitanti). Se non rappresenta uno spreco ed un costo inutile della politica questo fatto, non so quali altri possono essere individuati. propongo di modificare l'articolo del testo unico degli enti locali relativo ai consigli di circoscrizione e di limitarne la possibilità di istituzione solo nei Comuni con più di 300.000 abitanti. D'altro canto questo corrisponde pure alla logica in cui furono istituiti i consigli di circoscrizione, che rispondevano all'esigenza di articolare forme di decentramento nei grandi Comuni, nelle aree metropolitane, nei Comuni capoluogo di Regione; possibilità in modo indiscriminato con i risultati che ho poc'anzi ricordato. Ecco perché insisto per l'approvazione di questo emendamento, che certamente può rappresentare un contributo non marginale alla riduzione dei costi della politica.

avevamo ragione ieri quando sostenevamo che c'erano seri problemi di copertura del famoso emendamento 3.2000.

perché il Governo sulla scorta dell'intervento suo e nostro ha dovuto correggere la sua impostazione iniziale, tant'è vero che questa volta l'emendamento si fonda sull'allegato 7 della Ragioneria generale. Direi, dunque - non uso mai parole roboanti - che questo è uno smentirsi clamoro del Governo. Ci aveva provato; non ci è riuscito. Questo è tutto. Naturalmente se fosse soltanto un gioco tattico, sarebbe degno di una squisita discussione tra il sottosegretario Sartor, noi ed altri. In verità, queste cose sono il segno di una finanziaria che continua ad essere sempre più scoperta e cercherò adesso di dimostrare perché. In ogni caso, il Governo questa volta ha dovuto coprire l'emendamento dei *ticket* e non per cifre poco significative. Questo emendamento dice esattamente che per il 2008, che è l'anno che ci importava, il Governo ha dovuto attingere ben 97 milioni di euro direttamente dalle tabelle, 200 milioni di euro dalle manutenzioni e 447 milioni di euro per gli oneri del cofinanziamento delle opere dei Comuni. Si tratta di cifre assai significative e, quando si diceva che era pesante la scopertura di quell'emendamento, l'opposizione aveva ragione e la sua ragione gli viene dall'interlocutore autorevole che è il Governo.

non l'opposizione, ma un organismo autorevolissimo come l'Unione Europea certifica ormai che per il 2008 l'aumento del PIL è minore di quello previsto: nel DPEF - lo ricordo - era previsto all'1,7

della crescita del prodotto interno lordo crea un'ulteriore scopertura. Non c'è dubbio su questo. Calibrata sull'1,5 della Nota di aggiornamento

Non sembri, signor Presidente, lo 0,1 per cento del PIL qualche spicciolo; è qualcosa che cifra 1,5 miliardi di euro. Le scoperture sono, quindi, Questo ad ammettere che si mantenga il *trend* dell'1,4 per cento. Se ciò dovesse diminuire, è evidente che questa finanziaria nell'anno prossimo porterà una considerevole scoperturae dunque la possibilità di nuove tasse per gli italiani. Signor Sottosegretario,

si muove però in un quadro ancora abbastanza indefinito, perché quando parliamo dei 200 milioni delle manutenzioni lei sa meglio di me che si tratta di cifre che poi vedremo se si realizzeranno o meno. Se questi risparmi si trovano in un contesto di crescita minore, è molto più difficile ottenerli. Quindi, non soltanto la scopertura generale della finanziaria aumenta, ma anche questo emendamento riferito ai soli *ticket*, *ticket*, in un contesto declinante dell'aumento del prodotto interno lordo, presenterà margini di scopertura. Viassicuro, signor Presidente e signor Sottosegretario, che già in sede di assestamento saremo attenti a verificare se queste coperture si sono esattamente realizzate o meno e di quanto non si realizzano in ragione di ciò che ho detto, cioè sia della crescita declinante, sia della non certezza della riduzione di alcune di queste grandezze. Infine, nel merito, scherzando scherzando scherzando, abbiamo di nuovo inciso sull'unica cosasu cui non si deve incidere, la spesa per investimenti, perché - lo diciamo sempre tutti, maggioranza ed opposizione - è la spesa corrente che dobbiamo ridurre, non la spesa per investimenti. Noi invece per coprire spesa corrente utilizziamo spesa per investimenti per la parte maggiore, perché l'esclusione dal Patto di stabilità delle spese in conto capitale sostenute per interventi cofinanziati dall'Unione Europea riporta di nuovo una dura riduzione alla spesa per investimenti e questo naturalmente non fa bene, si riduce la spesa per investimenti per finanziare spesa corrente; un altro degli elementi che sottopongo all'attenzione della Presidenza e del Governo per chiedere che cosa stiamo facendo.

capacità di spesa per il conto capitale, che invece è ciò che serve in Italia. Infatti, o è vero che in Italia servono infrastrutture e investimenti o è vero che ci si muove in un contesto che si avvia al federalismo e quindi nella spesa per investimenti è importante quella degli enti locali, oppure non è vero, e allora dite bugie. Ma se fosse vero - ed è vero per molti Comuni ed enti locali - l'emendamento in esame li penalizza fortemente. Non solo,

per questa parte si tratta di 440 milioni - al conto corrente che è stato distribuito in giro nel corso della finanziaria. Ripeto, non è uno sforzo sul piano tecnico; probabilmente è uno sforzo molto grave sul piano politico, perché

la maggioranza. Non si capisce perché mai rigorosi custodi, come amano definirsi, della spesa pubblica, come il ministro Padoa-Schioppa, finanziano spese di conto corrente con spese in conto capitale e in maniera così incerta, mentre il prodotto interno lordo declina.

durante il percorso del disegno di legge finanziaria nell'Aula del Senato, se le sue previsioni di copertura, tutte impostate sulle nuove entrate, sono ancora valide, in una

è irrituale, di imporre al Governo un'ulteriore riflessione sulla copertura di questo emendamento, che parte disgraziato in origine e arriva a conclusione con un esito veramente paradossale. Per eliminare un'ingiustizia, un *ticket* sbagliato e improvvido, viene utilizzata una modalità di copertura che penalizza le spese virtuose per gli investimenti e le

imposto, diciamo così, un supplemento di riflessione al Governo. Oggi questa copertura è tecnicamente ineccepibile, ma politicamente assurda.

dell'Assemblea, quando siamo giunti a questo punto, perché non si poteva più sostenere una situazione nella quale operavamo al di fuori delle regole regole di buona amministrazione dello Stato. Avevamo quindi seri problemi dal punto di vista della

la nuova copertura trovata non è irrilevante al fine degli equilibri finanziari del Paese.

occorrerà aumentare il prelievo o tagliare altre spese. La copertura così determinata non avrà nessun livello di affidabilità

le censure e le preoccupazioni manifestate da parte dell'opposizione erano state confermate da un dato oggettivo.

I soldi, se disponibili, andavano indirizzati subito su questo tipo di intervento e non su altri tipi di interventi microsettoriali a pioggia, che sono serviti soltanto per consentire alla Commissione bilancio di esaurire i suoi lavori senza mal di pancia all'interno della maggioranza. Questo è un fatto politico che io ritengo di dover denunziare in quest'Aula,

intervengo solo per dire che su questo argomento di violento significato antimeridionale l'UDC ha già parlato abbondantemente e sono lieto che ora siano molti i colleghi

Adesso sono stati trovati i soldi a danno degli enti locali e, a nostro giudizio, questa copertura potrebbe anche essere insufficiente. Attendiamo il parere del Presidente della Repubblica sulla sua regolarità.

«Proporre, in Italia ed in qualche altro Paese di Europa, di abolire il "prefetto" sembra stravaganza degna di manicomio. Istituzione veneranda, venuta a noi dalla notte dei tempi L'Italia nuova, preoccupata di rinsaldare le *membra disiecta* degli antichi ex-Stati in un corpo unico, immaginò che il federalismo fosse il nemico ed estese il sistema prefettizio anche a quelle parti Si credette d'instaurare libertà e democrazia e si foggiò lo strumento della dittatura». Queste parole, signor Presidente, le prendo a prestito dal primo presidente della Repubblica italiana, Luigi Einaudi, che nel 1944, firmandosi Junius, come spesso faceva, ha parlato di come sia terribilmente sbagliato pensare di coniugare democrazia e prefetti. Noi, caro Presidente, siamo profondamente scontenti e addirittura offesi che esistano ancora delle cariche in Italia che impongono di chiamare "eccellenza" un dipendente dello Stato, che nelle cerimonie parla per ultimo, mettendo sotto di sé tutte le persone che vengono democraticamente elette a rappresentare i cittadini nel territorio, dai sindaci ai Presidenti di Provincia, ai Presidenti di Regione. Noi dubitiamo fortemente, signor Presidente e colleghi, che una democrazia possa avere ancora questo tipo di carica, perché da una parte dà ai cittadini il diritto di eleggere la propria rappresentanza e dall'altra il Governo centrale manda sui territori dei dipendenti che non hanno nessun altro merito, se non quello di essere la *longa manus* del Ministero e del centralismo, come se da viceré supplissero al potere di un sindaco che fa parlare in consiglio comunale il segretario e il segretario illustra quali sono i programmi e persegue coloro che non seguono i suoi programmi. Questo, oltre ad essere assolutamente contro la dignità di ogni cittadino, non può assolutamente permettere la crescita di una classe politica che possa finalmente portarci alla libertà e al federalismo. Sprono pertanto i colleghi, di qualsiasi parte siano, a smetterla di essere succubi delle "eccellenze". Chiedo

parere contrario

come viene chiesto da molte associazioni dell'ambiente cattolico. Immagino che non sarà neanche questo il momento e che rimanderete a miglior data.

Presidente, colleghi, prendo la parola per manifestare il profondo dissenso dei Popolari-Udeur sulla disposizione introdotta in Commissione che prevede l'istituzione del registro speciale dei simboli e dei contrassegni di partito e la relativa disciplina. A nostro avviso, l'introduzione di questa norma nel disegno di legge in esame rappresenta un'evidente forzatura per la mancata corrispondenza della stessa rispetto ai contenuti propri della legge finanziaria. L'articolo 11, comma 3, lettera *i*-bis) della legge n. 468 del 1978 (legge di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), infatti, annovera tra i suddetti contenuti le norme che comportano aumenti o riduzioni di spesa, con l'esclusione di quelle di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, come quella contenuta proprio nell'articolo 18-*bis*. La necessaria delimitazione dei contenuti della manovra economica è un'esigenza espressa in più di un'occasione anche dal Capo dello Stato per porre fine all'invalsa e scorretta prassi della finanziaria intesa quale contenitore *omnibus*. Nell'attesa di un'indispensabile riforma delle norme di legge e regolamentari che presiedono alla definizione del bilancio dello Stato, la verifica dei contenuti e le relative decisioni di buon senso sono ora rimesse agli organi competenti delle Camere ed in particolare alla Presidenza. Pertanto, la proposta che i Popolari-Udeur intendono sottoporre all'Assemblea è quella di procedere allo stralcio della norma in questione proprio a causa dell'assoluta estraneità della stessa rispetto alla legge finanziaria. A sostegno di questa affermazione, è l'attuale collocazione della normativa vigente, contenuta proprio nelle leggi relative alle varie consultazioni elettorali: l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati; l'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 recante norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario; l'articolo 11 della legge n. 18 del 1979 relativa all'elezione dei membri del Parlamento europeo, e così via dicendo. Certamente la nostra intenzione non è quella di chiudere un confronto sulla disciplina dei

su un tema delicato che presenta seri risvolti di ordine costituzionale, andando a toccare i princìpi della nostra democrazia rappresentativa. Un confronto ben diverso da quello svolto dalla Commissione

si celino movimenti oscuri di partiti che vogliono assicurarsi per legge posizioni di esclusività a discapito di altri. Chiedo, pertanto, l'accoglimento della proposta di stralcio in oggetto.

non avrebbe a monte dovuto entrare in una finanziaria, trattandosi di un tema estremamente delicato quale quello dell'utilizzazione dei simboli dei partiti e l'utilizzabilità nei momenti elettorali; l'avrei vista meglio in un testo di riforma elettorale, ordinamentale e non di carattere economico. Devo confessarle il mio stupore quando ho trovato tale testo introdotto nella manovra. Però l'abbiamo, siamo siamo chiamati a discuterne e vorrei evidenziare all'Aula come l'argomento sia estremamente e politicamente rilevante e delicato.

quella di risolvere in maniera giuridica e normativa il problema della concorrenza, dell'abuso di un simbolo similare e, quindi, della confusione

pone vincoli all'utilizzazione del simbolo in relazione alla presenza di quel movimento in Parlamento. Allora, signor Presidente, sono due tematiche estremamente delicate che andrebbero meglio integrate l'una con l'altra perché sono portatrici, a mio avviso, di due temi completamente diversi. Ripeto: il primo punto è condivisibile; l'altro andrebbe approfondito meglio perché, addirittura, la norma prevede

dell'utilizzazione del simbolo, perché in relazione a cosa dice il Regolamento della Camera e cosa il Regolamento del Senato in funzione del numero minimo perché possa essere rappresentato, è come se dessimo una delega ad altri.

e i colleghi di concedersi un momento di riflessione per una migliore elaborazione del testo perché in questo modo, così come è formulato, presenta dubbi secondo me anche di palese costituzionalità. Noi non ci sottrarremo al voto e dall'assumere le nostre responsabilità, però, premesso che si tratta di un tema che era meglio non trovare in finanziaria, riteniamo che uno sforzo collegiale da parte di tutti noi, maggioranza e opposizione, per poter riuscire a scrivere una norma, come si suol dire, a quattro mani, obbedirebbe alle regole di trasparenza della politica che i cittadini ci chiedono. proposta di stralcio illustrata dal senatore Barbato, ma la richiesta di accantonamento, avanzata dal presidente Schifani, essendo sull'ordine delle votazioni, ha la precedenza. Il Presidente,

17 e per altri emendamenti, si è ritenuto di accantonare un articolo o un emendamento, non vedo perché in questa circostanza non si possa accantonare l'emendamento un dibattito all'interno dell'Aula. Mi parrebbe una scelta di buonsenso, in sintonia con quanto è stato fatto fino ad ora. Devo aggiungere che io sottoscrivo completamente ciò che ha testè detto il collega Schifani, quindi una decisione che mi pare si possa prendere tranquillamente, come già capitato per articoli precedenti.

avrei preferito ascoltarla prima, la decisione che ho preso mi pare la più saggia, avendo ascoltato l'orientamento dei Gruppi. Passiamo quindi alla discussione sulla richiesta di accantonamento formalizzata dal senatore Schifani.

mentre invece siamo nella fase dell'accantonamento. Comunque, non ho difficoltà, se non per la diversità di vedute che a volte si registra all'interno del Gruppo che ci ospita, rappresentando io, come tutti sanno, l'Unione democratica. voglio dire con grande chiarezza, rispetto all'articolo 18-*bis* che è al nostro esame, che comprendo le ragioni profonde che hanno indotto i presentatori dell'articolo a prospettare al Senato una soluzione come quella nello stesso contenuta. Tuttavia, al di là delle ragioni non scritte (che possono essere comprese), noi abbiamo l'obbligo di misurarci con un testo

e come tutte le norme ordinamentali non ha alcun diritto di accesso in una legge finanziaria. Basterebbe, per fugare ogni dubbio, scorrere anche superficialmente il testo delle novelle introdotte in Commissione bilancio che gli Uffici, con la solita grande disponibilità e professionalità, hanno predisposto per cogliere (con il garbo solito agli Uffici), fra le righe, l'annotazione che siamo al cospetto di una norma che non avrebbe diritto di cittadinanza formale all'interno della materia che stiamo trattando. Ma è impresentabile solo perché è una norma ordinamentale? No, sarebbe poca cosa. È impresentabile perché siamo al cospetto di una materia tipicamente elettorale e quindi sensibile, che non può assolutamente essere trattata in maniera così superficiale come inevitabilmente, con l'inclusione all'interno di un articolo della legge finanziaria, accadrà. Ed ancora, signor Presidente, è impresentabile perché si tratta di una norma fotografia. Invito i colleghi che non l'hanno fatto a leggere l'articolo 18-bis, che ci tocca

anche sulla base di un precetto costituzionale, che non mi risulta essere stato soppresso, attendono ma aspirano, vogliono mettere in campo delle iniziative politiche. È incostituzionale, ancora, perché c'è una limitazione assoluta dei diritti dei singoli a partecipare e dei diritti delle associazioni partitiche perché è una norma protezionistica di una specie dell'esistente. Invitavo i colleghi a leggere la norma, perché è strutturata in maniera molto semplice:

C'è un assioma, signor Presidente, di questo tipo: chi oggi è in Parlamento e ha un Gruppo può depositare un simbolo (e questa sarebbe poca cosa), può depositare una denominazione precisa (e questo è un argine che diventa invalicabile e un confine insopportabile per la democrazia)

"democratico", "socialista" o tutti quegli altri termini che appartengono storicamente alla cultura politica italiana. Signor Presidente, la cosa più assurda è che all'interno di questo percorso ad ostacoli, che vuole tutelare soltanto l'esistente, c'è anche una limitazione che collide con il buon senso, perché prevede che siano autorizzati a depositare i simboli coloro i quali hanno un Gruppo adesso

di voler fare questa cosa un mese e mezzo fa. Come è possibile immaginare che un diritto indisponibile, come la possibilità di concedere di fare politica a chi ritiene di organizzarsi in un partito, in un movimento, in una associazione,

ha depositato il simbolo potrà autorizzare gli altri: ci si rende conto di come quelli che verranno domani, per poter fare politica utilizzando una parte di simbolo o di denominazione, dovranno soggiacere alle decisioni, alle pressioni o ai ricatti di quelli che già sono dentro? Signor Presidente, questo non solo per le elezioni politiche sarebbe poca cosa, ma anche per le elezioni amministrative, perché siffatto meccanismo a cascata - lo ripeto - si applica anche alle elezioni amministrative. non c'è problema rispetto alla violazione del Regolamento, la violazione della Costituzione è enorme, ma - signor Presidente, la affido a lei - la violazione del buonsenso è assolutamente insopportabile. Questa norma collide contro tutti i principi di ragionevolezza che un Parlamento civile come il nostro non può tollerare in maniera assoluta.

che vuole presentare simboli consimili nelle prossime - per qualcuno immediate - elezioni per mettere all'incasso l'immagine di qualcosa che è nella testa della gente, ma che non gli appartiene?

questo articolo - ringrazio il relatore per averlo presentato - solleva la problematica che, come vedete, ha avuto subito i suoi effetti: questa mattina, con centinaia di migliaia di euro di chissà chi, sono state comprate varie pagine di giornali costosissime per dire delle balle.

tante cose che non avrebbero dovuto essere presentate nella finanziaria, perché non c'entrano nulla con fattispecie eguali a quella in questione, come ad esempio il dimezzamento del numero dei consiglieri comunali? Quella non è materia elettorale, visto che si dimezzano i Consigli comunali d'Italia? Allora, perché protesta per questa norma e non per quella? Anche lei ha un secondo pensiero? L'esigenza di spianarsi la strada per fare qualcosa di simile a quello che c'è? c'è? Presidente, questa è una cosa realmente seria che, in qualche modo, mette in pericolo la Costituzione. Concludo dicendo ai più eminenti - io non sono un eminente giurista, ma una persona semplice che capisce e vorrei che capiste anche voi che siete tanto eminenti - che qui dentro sono presenti dieci Gruppi parlamentari, forse

dei DS, di Alleanza Nazionale o della Democrazia Cristiana perché, se non si è d'accordo con questo, allora si è tutti nell'imbroglio e nella confusione. Soltanto questo volevamo dire e dimostrare e vorremmo, votando mercoledì su questo

da tutti i membri della stessa, ad eccezione del rappresentante dell'Udeur. Vorrei ringraziare sia il relatore che il Governo che si erano rimessi al voto della Commissione, proprio perché stiamo trattando una materia che è

alcune motivazioni e sono contento di farlo prima che il Governo e il relatore esprimano il Presidente, noi siamo perché questa materia venga accantonata. Se è vero che ci sono motivi che potrebbero giustificare il miglioramento della norma, l'accantonamento serve a questo. Perché abbiamo proposto questa norma? Intanto noi riteniamo che questa sia una norma di trasparenza e di moralizzazione del sistema politico italiano. Abbiamo proposto l'istituzione, presso presso il Ministero dell'interno, di un Registro speciale per la tutela dei simboli e dei contrassegni di partito. Per quale motivo bisogna tutelare,

ci sono sentenze che prevedono riammissione di simboli e altre che prevedono la revoca di simboli quando la campagna elettorale è già iniziata, quindi, intervenendo in modo distorto e sbagliato sulla stessa campagna elettorale,

sia per quelle politiche, ad eccezione delle elezioni per il Parlamento europeo, con il sistema maggioritario. È diventata prassi nel Paese - ed è questo l'elemento di moralità

quei voti sufficienti per vincere, perché con questo sistema basta un voto in più per vincere e prendere il premio di maggioranza, come è successo del resto in alcune competizioni Quindi, questa è una forma di moralizzazione, per avere la garanzia che non possano essere utilizzati simboli simili o a volte persino uguali a simboli già presentati; ripeto, è una forma di moralizzazione.

fase in cui si va da un sistema ad un altro. Ci sono forze politiche che si stanno aggregando, forze politiche che si mettono assieme formando nuovi soggetti politici; questo processo produce aggregazioni e, nello stesso tempo, disarticolazioni. Ci sono state piccole scissioni; ci sono, anche in questo ramo del Parlamento,

in modo distorto nella competizione elettorale, laddove i cittadini hanno il diritto di esprimersi con tutte le informazioni, con tutta la chiarezza e con tutta la trasparenza. È questo il motivo vero

Nel merito della questione, condivido totalmente le considerazioni svolte dal collega Ripamonti: siamo in presenza di una disposizione legislativa che tende alla trasparenza e alla moralità del procedimento elettorale. Questo è il dato di fondo.

di una norma moralizzatrice e che consente maggiore trasparenza, in una fase delicatissima della nostra vita democratica, parlamentare e rappresentativa. Da questo punto di vista, l'UDC è favorevole alla proposta che il Presidente ha avanzato di votare, per ragioni

Un Paese forte, rispetto a problemi oggettivi che pure esistono e sono stati citati, non ricorre alla forza di chi è nel Palazzo

Mi sembra, invece, che i proprietari del Palazzo facciano di tutto per studiare una nuova legge elettorale "Erode", di modo che «chi è dentro è dentro, e chi è fuori è fuori» e non possono nascere altre formazioni politiche in grado di mettere in discussione questo sistema di potere.

Presidente, non è consueto, ma mi consenta innanzitutto di ringraziarla per aver fatto parlare i senatori anche se questo mi costa trenta secondi; però, che lei abbia preso una decisione saggia. Tenterò di contenere al massimo i miei argomenti, ma parlo anche a nome di una forza politica che nasce domani e rischia di morire dopodomani. Questo è inaccettabile lo dico con tutta la disponibilità alla discussione. Noi abbiamo tentato di seguire con coscienza i lavori della finanziaria;

non ce ne siamo accorti, evidentemente, per il lavoro, non sto dicendo per malafede. Presidente, si può mettere la democrazia nella legge finanziaria? La Commissione affari costituzionali non deve discutere questo? Credo che sia una questione importante, seria. Non voglio ripetere l'argomento del senatore Manzione: io le dico che sono favorevole allo stralcio. in tre e vi è una discussione in corso - probabilmente non parteciperemo alla votazione sull'accantonamento unicamente per una forma di rispetto per i colleghi e soprattutto per il collega che l'ha proposta, il presidente Schifani, perché non vogliamo arrivare Però - Santo Cielo! - la leggiamo questa norma? Ma se la legislatura, nonostante la nostra e sicuramente la mia volontà, durerà fino al 2011 e si formeranno altri Gruppi parlamentari, non potranno partecipare alle elezioni perché qui c'è il limite dei 90 giorni? Ma chi l'ha scritta questa norma? Poniamo l'assurdo che non passino né lo stralcio, né l'accantonamento e che precludiamo a questo Parlamento di formare altri Gruppi parlamentari se no non si partecipa alle elezioni, e tutto questo nonostante non ci sia una legge che regolamenta i partiti.

mettiamo i 5.000 euro. Ne legga la motivazione: questi 5.000 euro che devono dare i partiti concorrono ai saldi di finanza pubblica, al recupero del disavanzo. Allora Allora non è vero che vogliamo ridurre i partiti! Li vogliamo aumentare, perché almeno lo Stato recupera risorse. Ma non è ridicolo tutto questo? Questo trucco non è ridicolo? saldi di finanza pubblica si recupera il *deficit* perché ogni partito versa 5.000 euro (quindi 50.000, se sono dieci, o 100.000, Dobbiamo quindi incentivare il numero dei partiti, non ridurlo, cioè, si fa il *referendum* senza aprire le urne: lo si fa qua, durante la finanziaria. Credo che questo sia uno scandalo, Presidente! Infine, visto che ho usato la parola "*referendum*",

Se voglio sottoporre a *referendum* questa norma, che dà soldi allo Stato - 5.000 sporchi euro! - come faccio, Presidente? Credo che lei abbia la potestà di dichiarare inammissibile l'emendamento, perché si tratta di una questione grave. Detto questo, per la lealtà che mi caratterizza verso la coalizione, che spero non mi voglia espellere, ci limiteremo a non partecipare al voto sulla proposta del senatore Schifani per rispetto verso il presidente Schifani, ma non ci chiedete di mettere la gola sulla ghigliottina!

Signor Presidente, onorevoli colleghi, trovo veramente avvilente, avvilente, mentre è aperto un ampio e interessante dibattito sulla finanziaria, parlare di materia che ha una sua esclusiva e preminente valenza elettorale. È un gravissimo *vulnus* alle funzioni proprie della Commissione affari costituzionali del Senato. Infatti, mentre la Commissione affari costituzionali del Senato si occupa di riforma elettorale, si interviene, in maniera maldestra, ammettendo nel testo della finanziaria un articolo, peraltro inserito in Commissione, che è un vero e proprio colpo di mano ed un attentato alla democrazia del nostro Paese, al libero esercizio del gioco politico perché quando, in questo modo, si provvede ad introdurre surrettiziamente norme di chiusura rispetto alla libera partecipazione ad una competizione elettorale, significa perpetuare le logiche vere di una casta parlamentare, di una simbologia che si esalta attraverso il connotato vetero-politico che impedisce anche la costruzione e la partecipazione di nuovi soggetti politici. Ecco perché rinnoviamo al Presidente del Senato di rinverdire la sua potestà, anche in altre circostanze espressa e manifestata. Rientra nelle sue proprie competenze dichiarare inammissibile l'articolo della finanziaria e riconsiderare il problema nel più ampio contesto riformatore in corso di ragionamento nella Commissione affari costituzionali del Senato. Questo lo dico perché la scorciatoia pericolosa che può intervenire in presenza di un atto di testardaggine ed anche di miopia politica significa preparare l'abbrivio ad una crisi della maggioranza con connotati e pulsioni di tipo partitocratico che impediscono un confronto serio e limpido tra i partiti, soggetti della stessa maggioranza. Quindi, come Popolari-Udeur, che il punto venga stralciato e diventi parte essenziale di un procedimento all'interno della Commissione affari costituzionali. *(Applausi

penso che potremmo essere tutti d'accordo con lo spirito che ha animato l'iniziativa del senatore Ripamonti e quella di tanti altri colleghi, cioè l'esigenza di avere una semplificazione nella registrazione dei simboli elettorali e di improntare ad una forte trasparenza e moralizzazione questo atto politico ed istituzionale, che ha un peso ed una rilevanza enormi nella vita democratica del nostro e di ciascun Paese. Penso, però, anche che possiamo essere tutti quanti d'accordo su una considerazione ovvia ed elementare, cioè che questa è una norma

Cari colleghi, non ne voglio fare una questione di lana caprina sull'ammissibilità di questo emendamento così rilevante ed importante. Però, secondo me, una riflessione che veniva poco fa accennata, se non sbaglio, da parte del senatore Schifani, non è priva di fondamento. Questa è una materia, data anche la specifica e particolare contingenza politica che vive il nostro Paese, di estrema delicatezza

di forze o movimenti politici rappresentati in uno dei due rami del Parlamento da un Gruppo parlamentare. Faccio loro notare che in primo luogo, come è del tutto il evidente, la legge demanda ai Regolamenti parlamentari di Camera e Senato

norma, così definita, crei una difficoltà pressoché insormontabile per nuove forze politiche a presentarsi con un determinato nuovo simbolo alle elezioni politiche. Per esempio, se dovessimo andare al voto domani mattina (la questione non riguarda soltanto piccole forze politiche), il nascente o nato Partito democratico non si potrebbe presentare alle elezioni con tale denominazione. In terzo luogo, la questione che va sottolineata è molto semplice. Signor Presidente, noi siamo nel Senato della Repubblica. Si dà il caso nel Senato della Repubblica. Si dà il caso che nella Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica sia in corso di discussione la modifica della legge elettorale.

Questo lo dico, signor Presidente, perché mi sembra del tutto congruo che questa materia, ripeto, così rilevante e delicata, non sia affrontata nel contesto di una già travagliata legge finanziaria,

di illustrare bene all'Assemblea la situazione, perché in molti colleghi penso ci sia un po' di confusione.

D'altro canto, noi la condividiamo nella *ratio* perché ci sono troppe «liste patacca» durante le elezioni e questa è una piaga assolutamente da eliminare.

Presidente, durante il dibattito su questa finanziaria abbiamo assistito

e questo non è capitato una volta sola, ma più volte in questi tre giorni di dibattito e di votazioni. Ora c'è questo

Avevamo tentato di trovare una soluzione, chiedendone l'accantonamento, in modo da poter avere due o tre giorni di tempo per vedere se trovavamo un punto d'incontro su un articolo che certamente non c'entra assolutamente con la finanziaria. Nella precedente legislatura, il Presidente della Repubblica non avrebbe mai firmato

il provvedimento, che però è stata ammessa e votata in Commissione e portata in Aula, ora si chiede lo stralcio. Di fronte a questo atteggiamento, francamente non ce la sentiamo nemmeno di esprimere un voto:

questo articolo che oggi, dopo averlo proposto, chiede che non sia più discusso e che venga stralciato dalla finanziaria stessa. Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare il senatore Ripamonti per aver presentato questo emendamento. Nella storia di questo Parlamento, il senatore Ripamonti resta il primo che ha osato sfidare la casta, quella vera, che è quella che siede qui, viene eletta con liste, fa politica, ma si è rifiutata (dal 1946 ad oggi) di normare l'unica associazione non riconosciuta di rilevanza costituzionale che non ha alcuna norma che la regoli: i partiti politici. Dopodiché, la casta è brava e quindi oratori brillanti ci hanno spiegato che questa norma (che non era null'altro che una norma anticontraffazione applicata alla politica) diventava una norma liberticida solo perché istituiva un registro - si badi bene - che non impediva al cittadino di presentare un simbolo

senatore Ripamonti potrebbe fermarlo. L'emendamento Ripamonti, votato all'unanimità dai membri non ancora ricattati della Commissione, quell'emendamento, votato unanimemente da tutte e due le coalizioni, si limitava semplicemente a impedire che un cittadino che intendesse fondare un partito potesse rubare il simbolo ad un partito già presente in Parlamento. Questo era tutto. Ma la casta, rappresentata al massimo livello da alcuni oratori, ha stabilito che questa norma non si deve fare. Cosa resta, per difendersi? Signor Presidente del Senato, io guardo da quella parte e vedo uomini che non sono certamente sostenitori della mia linea: vedo il presidente Colombo e il presidente Scalfaro, con cui tante polemiche abbiamo avuto in questi anni. Mi permetta, signor Presidente, ma se io leggo sul «Corriere della Sera» che il partito che loro hanno servito per una vita esiste e presenta il simbolo storico addirittura sottraendolo ad un partito mio alleato ma non sempre amichevole, come l'UDC, e una denominazione come quella di questo Gruppo parlamentare; se penso che le elezioni politiche sono state vinte da una Lega fasulla, che ha rubato 80.000 voti alla Lega Nord e ha portato la sinistra al Governo; se penso che noi stavamo per vincerle battendo la Lega fasulla con un partito dei Verdi fasullo che la coalizione di Berlusconi aveva associato a sé, penso: ma, ragazzi, io Forcella l'ho frequentata, perché prima di andare all'università ci andavo a comprare qualcosa a buon mercato, però, ho l'impressione che questa è diventata la Forcella d'Italia, perché qui siamo di fronte ad un tentativo di perpetuare l'imbroglio e voi vi trincerate nei colloqui privati dietro il ricatto di Mastella. Allora, domando al ministro Mastella: ma quale diritto rivendica alla sua maggioranza, di rubare il simbolo a Casini? Che passiamo da Forcella

Colleghi senatori, ci stiamo rendendo complici di un imbroglio, che lasciamo tutto a voi perché i senatori della Democrazia Cristiana abbandonano l'Aula

semplice. Già all'inizio del mio precedente intervento, che era procedurale, ho dichiarato che se fossimo passati al merito avrei affrontato il merito, ho anticipato soltanto l'apprezzamento per l'iniziativa del collega Ripamonti, ritenendola moralizzatrice e trasparente. Confermo questa idea: le affermazioni dei colleghi Rotondi e Matteoli rendono evidente che si trattava e si tratta di una norma moralizzatrice e trasparente. Per queste ragioni, non ci interessa l'esito dello voto: abbiamo votato a favore dell'accantonamento e siamo stati sconfitti, voteremo contro lo stralcio e saremo sconfitti,

tra due tematiche scritte non perfettamente, seppur portatrici di esigenze sulle quali si poteva anche legiferare. Ritenevo prevalente e più degna di attenzione la tematica

similari ad altri presenti e si potesse indurre l'elettore in errore in relazione al voto che esprimeva chiamato in cabina elettorale. Questo non è accaduto ci troviamo dinanzi ad una norma che, così com'è scritta, effettivamente contiene dei punti meritevoli di modifica sostanziale e mi riferisco, in particolar modo, alla seconda parte. Così non Così non è stato, prendiamo atto della volontà dell'Aula, ma anche noi non ce la sentiamo di partecipare al voto su una scelta della quale la maggioranza si deve assumere l'intera responsabilità. La maggioranza ha bocciato la nostra richiesta di approfondimento per migliorare la norma, la maggioranza è chiamata quindi a prendere atto pubblicamente della sua volontà di tornare indietro su una scelta che aveva portato avanti in Commissione.

impegnare più di un'ora di tempo per il dibattito su un argomento che meritava sicuramente notevole attenzione in ambito diverso rispetto a quello della manovra

situazioni trasversali che la portano alla paralisi (probabilmente qualche alleato essenziale che magari alza la voce per ottenere lo stralcio; lo abbiamo capito abbondantemente

Signor Presidente, sinceramente noi siamo ragazzi, ma non ragazzini: non cadiamo in certe trappole; capiamo bene le cose. Questo testo è improponibile e, quindi, noi coerentemente voteremo per lo stralcio. Se l'UDC, come tutta la Casa delle Libertà, fosse uscita e non avesse partecipato al voto, anche noi

C'è un *deficit* nell'ordinamento giuridico del nostro Paese che riguarda anzitutto la disciplina dei partiti politici; c'è un *deficit* che riguarda la materia delle elezioni primarie; c'è un *deficit* che riguarda la questione relativa ai simboli dei partiti. Proprio per tale ragione sono state depositate in questa legislatura ed in questo ramo del Parlamento numerose proposte di legge da parte di colleghi. La Commissione, che ho l'onore di presiedere, ha avviato l'esame - ascoltando, tra l'altro, una relazione molto apprezzata dal punto di vista anche tecnico del collega Fisichella che riguarda alcuni di questi aspetti - che credo sia necessario e doveroso che la Commissione riprenda subito dopo la legge finanziaria, in concomitanza naturalmente con l'esame anche della riforma della legge elettorale.

volevo rispondere a una sconnessione lessicale - spero - del collega Rotondi, come ex ragazzo democristiano per quanto mi riguarda.

5.000 sporchi euro non possono legittimare il diritto di intrapresa di qualsiasi cittadino italiano che voglia realizzare un consorzio di associazione per realizzare una forma di partito. Questa è la democrazia; credo che questo debba essere anche lo spunto

e per chiedere al Governo e al relatore un impegno preciso perché ci sia la possibilità di riprendere queste questioni in altra sede. Spero che ciò avvenga all'interno

È un tema che serve prima di tutto al popolo sovrano e agli elettori, perché quando si taroccano i simboli si fa danno alla democrazia. Vogliamo che questo tema venga risolto e ci dispiace che qualcuno in quest'Aula, per contrastare questa iniziativa, abbia persino detto che la stessa era finalizzata a impedire che altri potessero costituire altri partiti

sottolineato efficacemente dal senatore Ripamonti, ma lo rinvia ad altra sede, ovvero alla riforma della legge elettorale o ad altro provvedimento legislativo. Così stanno le cose e ci tenevo a precisarlo.

del costo di una patologia, quella della chirurgia della cataratta, che nel tempo è divenuta sempre più costosa a motivo del maggior costo dei materiali applicati per questa patologia. Probabilmente oggi non sarà possibile risolvere questo argomento, ma la Ministro della salute, che è presente, vorrà prendere - occorrendo - buona nota perché nei tempi e modi dovuti, in altra sede, ma con solerzia, si possa favorevolmente accogliere questa proposta per consentire al Servizio sanitario nazionale di essere ristorato dei maggiori costi che si sono avuti nel corso dell'ultimo periodo.

Vorrei sottolineare ai colleghi che finalmente, in questo disegno di legge finanziaria, che ha visto solo emendamenti a favore di Comuni male amministrati e in soccorso dei disastri degli enti locali, si tratta di un emendamento che invece vuole premiare i Comuni che hanno ben utilizzato i finanziamenti governativi. Il "Programma Urban Italia", infatti, fu introdotto dalla legge finanziaria per il 2001, ed è stato puntualmente utilizzato dai Comuni beneficiari - sono 20 Comuni in tutta Italia, sparsi su tutto il territorio nazionale - che hanno usato i fondi, rendicontato fino all'ultimo centesimo quei fondi assegnati e trasformato il volto delle loro città. È chiaro che quell'intervento, a suo tempo integrativo di un finanziamento europeo, non fu esaustivo dello sforzo progettuale fatto da quei Comuni. Quindi, credo sia un segnale di attenzione integrare quel finanziamento, consentire a quei Comuni virtuosi di completare i loro interventi progettuali e quindi di definire il riassetto urbano delle loro città.

testé illustrata dal collega Turigliatto. Come lei sa e come sicuramente sanno tutti i colleghi, il prossimo vertice dei Paesi più industrializzati del mondo si svolgerà in Sardegna e, in particolare, nell'isola Mentre a Roma il Governo individua nel vice *premier* Rutelli il commissario incaricato di questo evento, relegando la Sardegna ad un ruolo del tutto secondario di comparsa, i sardi sognano

Pallaro di essere attento e così mi rivolgo ai senatori dell'emigrazione italiana nel mondo: proponiamo di fondare un grande museo italiano a Buenos Aires, che è la capitale dell'emigrazione italiana nel mondo.

Mi rivolgo ai senatori della sinistra antimperialista: in una storia ideale dell'antimperialismo in America latina questo è un momento cruciale. Cosa proponiamo di fare? Proponiamo di realizzare un museo italiano che sottolinei

con prestiti di opere che giacciono inutilizzate negli scantinati dei nostri musei - opere che spesso non sono garantite contro l'umidità, non hanno il controllo di temperatura, non hanno neanche gatti che le difendano contro i topi

perché questa sarebbe un'operazione esemplare, che dice il rilievo che il Paese dà al fenomeno dell'immigrazione. Invito caldamente a non giudicare questa proposta in un'ottica di parte, bensì a votarla come segno di italianità.

al fine di promuovere la cultura italiana nel mondo, si potrà ugualmente conseguire il medesimo risultato, magari in altra forma. In tal senso, solleciterei un ordine del giorno del senatore Buttiglione potrebbe affrontare e risolvere il problema, demandando al Governo la valutazione sull'opportunità e possibilità di realizzare tale obiettivo.

Intendiamoci: c'è già un museo internazionale dell'emigrazione a Buenos Aires, ed è il *Memorial de los Inmigrantes*, uno dei più importanti musei della emigrazione al mondo, e la direttrice del museo è stata invitata, dieci giorni fa, per una riflessione sull'istituzione a Roma, invece, di un museo dell'emigrazione italiana, cosa che dobbiamo alla diaspora italiana. Se invece il senatore

e la città di Buenos Aires o lo Stato argentino ci concederanno gratuitamente un immobile, nel quale utilizzando, in maniera credo positiva,

una operazione che si farà anche in altri Paesi - di pregustare la qualità delle opere d'arte italiane, per poi venire direttamente in Italia ad ammirarle ed è un'operazione che realizzeremo a costo a zero. *(UDC)*. Ricordo al Vice ministro che i contatti con il Governo argentino in tale materia furono iniziati sotto il Governo Berlusconi dall'allora Ministro per i beni culturali e che il progetto, però, fino ad ora, non ha avuto nessun svolgimento. Ho atteso un anno ed ho pensato di intervenire in sede parlamentare per rimetterlo in cammino. La mia modesta opinione

argentino, propenso a metterlo a disposizione - ma vi sono lavori di ristrutturazione da fare su quell'immobile ed esistono comunque una serie di vicende connesse, le quali fanno ritenere opportuno il provvedere un adeguato stanziamento, altrimenti ho il sospetto

vorrei ricordare che il nostro Paese non ha ancora saputo o non ha ancora voluto fare chiarezza su quella che Amnesty International ha ha definito la più grave sospensione dei diritti civili nel nostro Paese, dopo la Seconda Guerra Mondiale. questo, penso che il nostro Paese non possa permettersi un nuovo G8. Quindi, voterò a favore dell'emendamento. Presidente, vorrei chiedere al collega Buttiglione, se me lo consente, di aggiungere la firma a questo emendamento e, in quanto vice presidente del Comitato per gli italiani all'estero,

Presidente, l'articolo 22 tratta dello sviluppo professionale delle Forze armate. Il comma 1 incrementa il fondo già esistente di 30 milioni. Con il nostro emendamento 22.5 proponiamo di destinare il 50 per cento di questo incremento per consentire ai volontari in ferma breve delle Forze armate con almeno tre anni di servizio, aventi tutti i requisiti previsti, di poter transitare nei ruoli di truppa del servizio permanente

per l'operatività quotidiana della forza di polizia più capillarmente diffusa sul territorio nazionale. Non credo che cadrà il Governo o si altererà il bilancio dello Stato se la funzionalità dei Carabinieri passa da 40 a 100 milioni di euro nel momento in cui l'intero comparto Viminale è interessato da un taglio di 840 milioni di euro. Più volte in questi giorni ci è stato detto che la sicurezza non è né di destra né di sinistra: il centro-sinistra ha l'occasione di dimostrarlo nei fatti con un voto favorevole a questo emendamento, sul quale chiedo la votazione

tanti altri incidenti, tanti altri episodi di altrettanta gravità e pericolosità sociale, ma finché sono accaduti al Nord non c'è stato un grande interesse. Volevamo rimarcarlo.

La legge finanziaria 2004 destina una somma di 120 milioni di euro per avviare (soltanto avviare) una riforma degli assetti del personale delle Forze di polizia in attesa da anni, il cosiddetto riordino. Le successive leggi finanziarie, inclusa quella del Governo Prodi lo scorso anno, quindi quella del 2007, hanno sempre confermato questo appostamento che poi non è stato utilizzato per una serie di ragioni, non ultima, un certo disaccordo tra le organizzazioni sindacali e le rappresentanze su come realizzare il riordino. Il disaccordo, tuttavia, non sul se, per cui se scompare questa posta dal bilancio, e l'emendamento punta invece a confermarla, è certo che il riordino non ci sarà È evidente che, una volta partito, poi va completato con risorse da appostare sulle successive finanziarie. Allora, prima del voto, chiedo che il Governo riveda il proprio parere per non essere in contraddizione con se stesso, perché nel 2007 ha mantenuto questa posta in bilancio, nell'ottobre del 2006 il vice ministro Minniti confermò in 1a e 4a Commissione che la posta c'era e che era intenzione del Governo in carica di realizzare il riordino e la stessa conferma c'è stata nel mese di ottobre 2007. se non vuole contrastare se stesso, il Governo non può che accogliere questo emendamento; se è necessario un approfondimento ulteriore per verificare se ciò che sto dicendo non è conforme al vero,

Mi rimetto al Governo. la forma tecnica attraverso la quale si vuole mantenere la somma stanziata negli anni precedenti per il riordino delle carriere. possibile e non è opportuno farlo in legge finanziaria in quanto si violerebbe una norma generale che limita le riassegnazioni. Posso assicurare che il Governo sta provvedendo a mantenere, come ha già fatto nello scorso anno, la cifra a suo tempo stanziata con provvedimento che riguarda il bilancio e non la legge finanziaria. Quindi, confermo l'intendimento del Quindi, confermo l'intendimento del Governo di mantenere lo stanziamento che è stato disposto negli anni passati e che, come giustamente ricordato, non è stato ancora utilizzato, però questo mantenimento non è opportuno che avvenga in legge finanziaria perché contrasterebbe con una norma generale che vieta la riassegnazione. La sostanza della proposta rimane accolta in forma diversa. PRESIDENTE. Se fosse un ordine giorno il Governo sarebbe favorevole?

per le Forze armate, e sull'articolo 22-*bis*, che tratta le misure a sostegno del personale operante in aree militari, sia io che il collega Ciccanti abbiamo votato a favore perché crediamo che il sostegno alle Forze armate e ai nostri militari all'estero non vada mai sottratto.

che due persone completamente travisate, si trovavano del tutto indisturbate, evidentemente dopo avere passato tutti i controlli, nell'area delle partenze internazionali dell'aeroporto di Malpensa. L'interrogazione acquisisce acquisisce ulteriore gravità per il fatto che porta all'attenzione del Governo, in quanto proprio in Commissione affari costituzionali abbiamo udito dal prefetto Cazzella che esiste un documento diffuso dal Ministero dell'interno in cui si esclude specificamente un tale tipo di vestiario - si intende la copertura totale del capo e del volto in qualunque situazione pubblica e, in particolare, di questo genere. Visto che il Governo ha ritenuto di dover emanare un decreto-legge sull'argomento della sicurezza, sarebbe bene che desse anche una chiara risposta ad un fatto precisamente documentato (con tanto di ora e circostanza e per il quale sarebbe facile trovare i responsabili) per sapere se girare in un luogo delicato per la sicurezza come un aeroporto internazionale sia teoricamente proibito dalla legge, ma di fatto consentito, e chi ha stabilito di prendere questa decisione. Presidente, la ringrazio moltissimo per avermi dato la parola: in omaggio al Regolamento che ci consente, al termine della seduta, di poterla richiedere. Il Regolamento ci offre anche la possibilità di sollecitare risposte del Governo ad interrogazioni. Ebbene, credo che sia questa la quarta o quinta volta che sollecito una

Sfortunatamente a seguito della sua scomparsa, della quale dal punto di vista umano ci dispiaciamo (anche se dopo la morte dei miei genitori quasi tutte le morti mi lasciano indifferente:

si è scatenata in un assalto non sulla memoria di Biagi o per parlare doverosamente della sua storia, ma in un vero e proprio assalto alla diligenza (vedi "Anno zero" ieri sera, senza contraddittorio,

si sia profuso in considerazioni - lui personalmente, lui il giornalista - sul famoso e cosiddetto «editto bulgaro», permettendosi di liquidare il *leader* di un partito di opposizione, l'*ex* Presidente del Consiglio, con parole irriguardose. È poi inutile parlare di Santoro, perché la sua storia è conosciuta a tutti.